Signora Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame pone in evidenza alcuni dati. Il saldo netto da finanziare fissato dalla legge di bilancio è di 32,7 miliardi di euro; con l'assestamento, il saldo netto da finanziare passa invece a 69,6 miliardi di euro. Il risparmio pubblico, che nella legge di bilancio in vigore ha valore positivo per 12,7 miliardi, peggiora di 32 miliardi e diventa negativo per 19,6 miliardi. L'avanzo primario passa da 48,5 miliardi a 8,5 miliardi, con un peggioramento penso che il Governo ascolterà con attenzione e conosca questi dati - di 40 miliardi di euro, interamente determinato dalle proposte contenute nel disegno di legge di assestamento. Questi dati, signora Presidente, evidenziano due enormi problemi, uno di forma ed uno di sostanza. Quello di forma si può riassumere nel fatto che la legge di assestamento non può disporre scelte discrezionali di spesa con un peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento. Infatti, questo disegno di legge di assestamento non registra soltanto le minori entrate determinate dall'andamento macroeconomico, ma dispone maggiori spese discrezionali per almeno un punto di prodotto interno lordo. Il secondo problema, quello di sostanza, nasce dal fatto che il Governo fa una manovra espansiva discrezionale per un punto di prodotto interno lordo, usando questo punto per incrementare la spesa pubblica così com'è, senza alcun ordine di priorità. Tutti sappiamo che una strategia meramente incrementale della spesa, lasciando l'ordine delle priorità attuali, è nemica della buona politica, in particolare di quella tesa al risanamento ed al rilancio dell'economia. Infine, una piccola annotazione già fatta rimarcare da altri colleghi: nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, si istituisce il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, con 9 miliardi di euro a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Nel decreto-legge n. 39 del 2009, all'articolo 14, da 2 a 4 miliardi di euro sono utilizzati per finanziare gli interventi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto attingendo dal Fondo strategico con risorse del FAS. Nell'assestamento il Fondo strategico a sostegno dell'economia reale non viene menzionato. Quindi, Quindi, signora Presidente, c'è una legge che istituisce quel Fondo e lo dota di 9 miliardi di euro, c'è una legge che copre su quel Fondo per 4 miliardi di euro il provvedimento sul terremoto, ma nel bilancio il Fondo non c'è e non c'è nemmeno adesso che è stato presentato l'assestamento.

Sorge una domanda: dove sono i soldi per il FAS? Signora Presidente, i dubbi e le incongruenze del disegno di legge al nostro esame ci portano a capire che il Governo non sta governando la crisi, ma ne viene governato.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, un anno fa, in occasione dell'esame dell'assestamento di bilancio per l'anno finanziario 2008, l'allora sottosegretario di Stato Vegas all'opposizione, che lamentava una sorta di inerzia rispetto a un periodo in cui già si avvisavano elementi di drammaticità economica e sociale e in cui venivano richiesti interventi maggiormente incisivi nella finanza pubblica, rispondeva che è natura dell'assestamento di bilancio quella di non modificare la legislazione in atto, essendo il Governo intervenuto varando, con una modalità sostanzialmente innovativa, a suo dire, una manovra anticipata e triennale in misura alquanto cospicua con il decreto-legge n. Quest'anno il provvedimento in esame - ci è stato detto e ripetuto in Commissione - è qualcosa di diverso e noi dell'Italia dei Valori spiegheremo le ragioni della nostra contrarietà, una contrarietà chiara e forte a questa diversità. Abbiamo già detto che questo provvedimento non si limita soltanto a evidenziare un peggioramento del saldo netto da finanziare di 36,8 miliardi, attribuibile in parte alla rilevante diminuzione delle entrate, in parte ad un aumento delle spese finali di 4,5 miliardi. Fa di più: con un aumento delle autorizzazioni di cassa, pari a circa 18 miliardi, e con un impatto sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione del tutto evidente acquista la caratteristica sostanziale di una manovra espansiva di cassa del bilancio dello Stato. In sostanza, com'è stato più volte ripetuto in quest'Aula, un nuovo bilancio. E allora noi dell'Italia dei Valori vogliamo considerarlo come tale, mettendo da parte ogni valutazione tecnico-giuridica sul quesito se i contenuti di discrezionalità possano collocarsi o meno all'interno della portata funzionale di tale provvedimento. Riteniamo infatti che in questo momento tali tecnicismi sarebbero non solo incomprensibili, ma forse del tutto indifferenti a una massa di persone che quotidianamente fa i conti individuali con la crisi, non solo e non tanto in termini di perdita di valore, ma di sopravvivenza, di dignità umana, di ruolo sociale, in quanto ha perso, sta perdendo o non riesce a trovare, per la prima volta, quel bene prioritario che è il lavoro. Questo provvedimento impone quindi a nostro avviso alcune considerazioni. La prima. Esso è la conferma di un irresponsabile e dannoso ritardo del Governo a riconoscere le dimensioni quantitative, la portata e le conseguenze della gravità della crisi. Troppo spesso ci siamo sentiti ripetere che il PIL e le esportazioni diminuiscono, ma meno che altrove; che l'occupazione scende, ma più lentamente che nei grandi Paesi industrializzati; il deficit e il debito ci sono, ma la loro crescita è meno veloce che negli altri Paesi. In Abruzzo le risorse mancano, ma - ci è stato detto - non capite la differenza tra competenza e cassa. E le colpe di chi alimenta un presunto catastrofismo sono sempre assegnate agli altri, all'opposizione e, quando non è colpa dell'opposizione, in particolare agli organismi internazionali, colpevoli di sfornare ogni giorno cifre allarmiste che poi, purtroppo, si rivelano realiste. L'OCSE è invitata a stare zitta; i commissari europei a non disturbare il lavoro del Governo; il governatore Draghi a non fare solo congetture. In realtà il Governo ha dimostrato di essere ben più impreparato alla crisi di quanto ha voluto far credere perché sa benissimo, visto che le regole della comunicazione non gli sono estranee, che il suo fastidio o le sue risposte stizzite non servono ad allontanarla, ma nascondono solo la verità e, con essa, il suo parziale immobilismo. Pochi mesi fa il Fondo monetario internazionale ha stilato una classifica dell'attivismo discrezionale dei Governi, perché non c'è dubbio che sui saldi di un bilancio pubblico influisce la situazione economica che si vive (se le cose vanno male calano le entrate e crescono le spese), ma influiscono anche le misure assunte dai Governi e dai Parlamenti. E se la prima fonte di peggioramento dei saldi opera da sola, la seconda è discrezionale. Bene, l'Italia è all'ultimo posto con un contributo, in termini comparativi, praticamente nullo. Nel novembre dello scorso anno la Commissione europea, prima, e il Consiglio europeo, poi, hanno riconosciuto la necessità di contrastare la recessione economica, concedendo ai Paesi della zona euro un più ampio margine di manovra dal lato della politica di bilancio. Di fronte a questi segnali, il Governo del nostro Paese ha perseverato, continuando per mesi una impostazione difensiva di una politica economica che si preoccupava più del giudizio dei mercati sull'affidabilità dei nostri titoli di stato che di un sostegno vero all'economia o, meglio, a quei tanti bisogni privi dei requisiti necessari per godere della protezione pubblica. La seconda considerazione è consequenziale alla prima: la prudenza e il presupposto rigore finanziario del Governo non si apprezzano in nessuno dei risultati di finanza pubblica, per cui, rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, peggiorano l'avanzo primario, il risparmio pubblico ed il ricorso al mercato e aumentano le spese correnti, riducendo la spesa in conto capitale, ossia il contrario di quanto dovrebbe avvenire. La logica adottata dal Governo è stata quella di porre rimedio alle urgenze imposte dalla congiuntura con interventi tampone, innescando solo ritardi e insicurezza e dando prova soltando di spregiudicatezza comunicativa, come nel caso della detassazione degli straordinari in un momento di forte flessione della domanda di lavoro, o gli appelli rivolti ad espandere i consumi privati, con una fortissima contrazione del reddito disponibile delle famiglie, o il confuso annuncio di incentivare l'ampliamento degli immobili o, *dulcis in fundo*, emblematica, la vicenda del FAS, che è stato progressivamente utilizzato come un fondo di riserva, una sorta di bancomat, per la copertura dei più diversi provvedimenti, per cui i maggiori investimenti annunciati a varie riprese dal Governo non sono altro che il riciclaggio di risorse già predisposte nella precedente legislatura.

è normale il calo del gettito e oltre quale misura è legittimo sospettare un'evasione fiscale in aumento? La Banca d'Italia ha notato che nel 2008 il gettito dell'IVA, che dovrebbe andare di pari passo con i consumi, è diminuito dell'1,5 per cento, mentre i consumi in valori monetari crescevano del 2,3 per cento. Può essere, come ci è stato risposto dal Governo, che i consumi nella crisi si siano spostati verso beni ad aliquota IVA più bassa, ma può anche essere, come pensiamo noi, che i contribuenti evadano di più a causa di alcune norme, come l'abolizione dell'elenco clienti-fornitori e la modifica profonda di misure antievasione introdotte nella passata legislatura e la cui eliminazione, più che una semplificazione, ha piuttosto garantito al Governo un maggiore consenso derivante dall'alleggerimento degli obblighi di determinate categorie di contribuenti. l'altra partita da definire è l'effettiva utilizzazione delle risorse individuate nel bilancio di assestamento per far fronte ai crediti arretrati vantati dalle imprese nei confronti dell'amministrazione pubblica. Così come resta da valutare la portata effettiva - lo faremo nella prossima settimana - dei meccanismi agevolativi sugli utili reinvestiti dalle imprese, contenuti nel decreto-legge n.

considerando che in questo periodo ogni giorno in Italia falliscono 30 imprese e che da indagini condotte emerge un dato non molto incoraggiante, ossia che l'incidenza delle società con attese di perdita è cresciuta al 23 per cento. Terza ed ultima considerazione: le cifre sono importanti nell'assestamento di bilancio quando portano misure concrete e riescono a frenare la paura e il dramma di chi perde il lavoro. Il Governo ha varato alcuni provvedimenti con limitate risorse finanziarie, ma ha anche ma ha anche segmentato ancora di più il sistema degli ammortizzatori sociali ed introdotto elementi di discrezionalità che avranno riflessi negativi. Come abbiamo più volte richiesto, agli ammortizzatori per estendere la cassa integrazione a tutti i lavoratori senza discriminazioni, per istituire una vera indennità di disoccupazione e per ampliare la tutela a tutte quelle forme di lavoro flessibile che sono state introdotte negli ultimi anni. Oggi che ci troviamo in piena recessione non sarebbe accettabile, non sarebbe onesto far ricadere tutto il peso su queste categorie di lavoratori. Poco più di un mese fa il Governo dichiarava che era riuscito a tenere in ordine i conti pubblici senza mettere le mani nelle tasche degli italiani. Contrariamente alle intenzioni annunciate, il deficit pubblico è salito ben oltre il massimo consentito dalle regole europee. E questo, se è comprensibile per gli effetti della crisi internazionale, lo è molto meno per un Paese come il nostro le cui misure anticrisi, come vantava il Ministro dell'economia, non hanno inciso e non dovevano incidere sui conti dello Stato perché spostavano fondi da un impiego all'altro. E sarebbe ancor meno comprensibile se lasciassimo indietro, senza aiuto, la tutela dei più deboli. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, la stabilizzazione dei conti pubblici o gli equilibri dei saldi netti da finanziare non possono più rappresentare un alibi per l'azione del Governo. Il Paese si attende non astratte e a volte saccenti lezioni di economia,

Di fronte ad una situazione oggettivamente drammatica, ieri abbiamo discettato - ad onor del vero la Lega non ha partecipato a questa dotta disquisizione - su

una presunta rinascita dell'evasione fiscale ed il fatto che la pressione fiscale resta

Ricordiamo che voi volevate dare la carta di credito a tutti, anche alla vecchietta, imponendo anche a lei di pagare interessi e commissioni per comprare il pane. Questo perché, secondo voi, non bisognava più usare la moneta contante.

Dietro questo ragionamento sull'evasione fiscale noi leggiamo due preoccupanti retropensieri. Il primo è il solito retropensiero secondo il quale chi ha la partita IVA è automaticamente un evasore.

miliardi del bilancio pubblico non li paghiamo mica noi con le tasse sulla nostra indennità, che ci paga comunque lo Stato, non li pagano mica i dipendenti pubblici, che i soldi li ricevono dallo Stato:

E continuare a pensare che chi ha la partita IVA sia automaticamente un evasore fiscale non vi porta da nessuna parte: vi allontana sempre più dal Paese reale.

Bisogna ridurre la spesa pubblica. Invece voi proponete il recupero dell'evasione fiscale. Ricomincia lo stesso spettacolo della scorsa legislatura: è impossibile, secondo voi, tagliare la spesa pubblica.

Vogliamo abolire le comunità montane, vogliamo tagliare una volta per tutte tutti gli enti e i carrozzoni inutili e voi, invece, volete rifinanziare le comunità montane.

Intanto basterebbe andare a leggere come si calcola la pressione fiscale: la pressione fiscale si calcola dividendo tutte le entrate derivanti da imposte e contributi per il PIL.

con tutte le difficoltà dei conti pubblici, di rimediare alle storture che voi negli ultimi due anni avete imposto. Ricordiamo il fuoco di fila di Visco, Prodi e Padoa-Schioppa: tolti gli ammortamenti anticipati, inaspriti gli studi di settore inserendo gli indici di normalità economica, la deducibilità degli interessi limitata,

E allora, come dovremmo approcciare - e qual è l'approccio della Lega Nord - una situazione difficile e complicata come questa? Prendiamo ad esempio come ci siamo comportati sull'assestamento: non abbiamo proposto maggiori spese o modifiche di spesa. Abbiamo proposto due ordini del giorno su due questioni importanti, ma non ce la siamo sentita di dire «spendiamo di più».

accettiamo l'impegno serio del Governo di fare tutto il possibile per garantire i fondi necessari per far funzionare questi servizi, ma nulla di più. Oggi non possiamo più pretendere di spremere ulteriormente il limone, perché e questo deve essere evidente sempre più a tutti - la situazione è talmente complicata che non possiamo più pensare di incrementare la spesa incrementando le entrate, tassando ancora di più i contribuenti.

che si esce da questa crisi complicata in un solo modo: tenendo in piedi il settore delle imprese (e quindi favorendo i nostri imprenditori), considerando i contribuenti non evasori ma contribuenti e il settore privato come quello che mantiene il sistema

spero e mi auguro che non sia solo colpa nostra! Anche questa storia prima o poi dovrà finire. Questo assestamento è davvero una brutta cosa. Noi l'avevamo detto l'anno scorso, quando furono discussi la finanziaria e il bilancio: di fronte ad una crisi come questa ci voleva e ci vuole più coraggio. Ci fu uno scontro vero l'anno scorso, tra due impostazioni diverse di bilancio: da una parte il Governo e il ministro Tremonti, a sostenere a spada tratta che bastava tenere sotto controllo i conti e le tasse e lasciare passare la buriana;

della crisi, in modo da riprendere il cammino dello sviluppo senza lasciarci alle spalle troppi morti, soprattutto tra le piccole e medie

Ci avete detto di no come sempre ed ora ci presentate la ricevuta fiscale di un conto che è una vergogna, un fallimento totale. Ci avevate promesso del culatello e ci date soltanto l'osso! Bisogna tenere i conti pubblici sotto controllo. Bene. Scopriamo le carte: i conti sono materia fredda ma implacabile. Il saldo di bilancio passa da 32,7 miliardi a 69,6, più del più del doppio, ed il debito crescerà di 2 punti, per aumentare l'anno prossimo di altri 10-12 punti e avvicinarsi al 120 per cento, come negli anni peggiori del Paese. Complimenti per chi voleva tenere i conti sotto controllo!

e l'anno prossimo sarà a meno 0,4, il peggior risultato del Paese dopo 18 anni. Complimenti anche in questo caso, visto che il vostro obiettivo era tenere i conti sotto controllo!

Ci si dice: ma c'è la crisi! Certo che c'è la crisi. Per il Presidente del Consiglio, a dire il vero, sembra di no, ma se gli obiettivi vostri erano quelli che ci avevate indicato, ora dovete prendere atto che è un fallimento quasi totale. I conti vanno male; il Paese purtroppo non bene. Il sistema regge ancora. Sì, regge ancora. Le famiglie tengono, o meglio, tengono i denti stretti cercano di resistere in questo momento, anche grazie al calo dei prodotti petroliferi e ad alcune misure (come gli ammortizzatori, l'intervento sulle banche, l'auto) che ci hanno aiutato ed aiutano le famiglie a traghettare oltre questo momento. Ma, come vi avevamo detto, non basta! Noi vi chiedevamo un punto di PIL, almeno un misero punto di PIL per sostenere l'economia e lo sviluppo; alcune risorse vere per i pagamenti della pubblica amministrazione; di derogare al Patto di stabilità per fare investimenti; di mettere un po' di denaro circolante nel Paese per sostenere le piccole e medie aziende nella ricerca, nell'innovazione, nella *green economy,* nell'internazionalizzazione del prodotto. Ci avete detto di no e oggi ci presentate un assestamento dove mettete 18 miliardi, oltre un punto di PIL che andrà ad incidere di nuovo sulla spesa, che sarà una maggiore spesa. Una manovra di bilancio nell'assestamento che peraltro è un'altra è un'altra vergogna dal punto di vista tecnico. Tutto questo per pagare i fornitori e forse anche la deroga al Patto di stabilità che state approvando in queste ore alla Camera. misure giuste; fate due di quelle cose che abbiamo chiesto noi, ma le fate dopo sei mesi, mettendo una pezza che rischia di essere peggiore del buco. Vergogna nella vergogna! Nell'assestamento mettete delle risorse che ancora non sono legge, come la deroga al Patto di stabilità, e non inserite non inserite invece quelle che dovreste mettere. Il decreto-legge n. 185 del 2008 vi obbliga ad iscrivere in bilancio il Fondo strategico per il Paese che voi avete quantificato in 9 miliardi, finanziato con i fondi FAS,

che, purtroppo per il Paese, rivela che a guidarlo oggi c'è una classe dirigente e un Governo incapaci di affrontare una crisi come questa, ma anche una classe dirigente e un Governo che dicono bugie e che sono incapaci di assumersi con coraggio responsabilità responsabilità vere ma oggi necessarie più che mai. Noi e con noi il Paese cominciamo però a chiederci quando questa sceneggiata finirà. Per il bene del Paese, ci auguriamo il prima possibile.

creando precedenti mai verificatisi nel nostro Paese. Ci vuole più serietà verso un Paese in difficoltà e più rispetto tra di noi e nei

di provvedimenti come il rendiconto e l'assestamento. Forse è più utile stare ai fatti ed alle previsioni,

Grazie. in prospettiva, con la riforma della normativa di contabilità già approvata dal Senato ed ora all'esame della Camera, il provvedimento di assestamento diventa un adempimento eventuale e non più necessario; sarà cioè un ulteriore tassello di quel riordino complessivo degli strumenti di finanza pubblica, di cui peraltro auspichiamo una sollecita approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento. Cosa voglio dire con questa premessa? l'assestamento, di per sé, nell'ambito degli strumenti di finanza pubblica, ha certamente degli elementi normativi che lo connotano ma è già presente agli occhi del legislatore la sua natura addirittura eventuale. Credo quindi che sia stato piuttosto inopportuno soffermarsi su questo. Ed allora, se questa è la situazione normativa, è evidente la scelta del Governo. In una situazione di crisi, non eccezionale, ma unica dal dopoguerra in poi, addirittura da 80 anni in poi, il Governo si trova nella necessità di dover calibrare i propri interventi in relazione all'evolversi della crisi. Lo hanno notato anche autorevoli commentatori di giornali. Invece di misure eclatanti o massicce, che peraltro la situazione dei nostri conti pubblici non consente, il Governo sceglie di emanare provvedimenti puntuali in relazione al concreto evolversi della crisi. Direi che si tratta di terapie mirate e non di carattere generico.

Prima di questo provvedimento - vado solo per esempi - il Governo si trova di fronte alla necessità di erogare liquidità nel sistema bancario...

allora, in quel caso, il Governo adotta i cosiddetti Tremonti *bond,* perché quella è la prima delle necessità e quello è stato ritenuto uno strumento efficace, come poi si sta rivelando.

contribuire alla risoluzione della crisi. Dunque, questo provvedimento si innesta in una visione di politica finanziaria ed economica che, nel contesto dell'attuale situazione dei conti pubblici, cerca di fronteggiare la crisi e di dare segnali efficaci, in particolare al mondo delle

valere sulla spesa corrente. Ciò è impossibile e, infatti, i saldi peggiorano per due ragioni evidenti: da una parte, per le minori entrate conseguenti alla contrazione della produzione e, dall'altra, per le maggiori spese, concernenti, tra l'altro, le misure per alleviare la crisi occupazionale (che mi pare siano un dovere del Governo, il quale peraltro lo ha particolarmente a cuore). Ecco perché

Il Governo sta continuando con le sue manovre e lo vedremo quando discuteremo il cosiddetto decreto anticrisi, che oggi è in fase di approvazione presso l'altro ramo del Parlamento. in esame ci sono delle misure anticipatorie, che si completeranno in un disegno unitario con il prossimo decreto. Come noto, una delle esigenze maggiori è in particolare lo sblocco degli investimenti degli enti locali. Nel disegno predispone 1,5 miliardi per poter coprire le deroghe al Patto di stabilità che vengono lì stabilite. non fa soltanto questo: nel provvedimento vi è anche un ulteriore stanziamento di 1,4 miliardi di euro per le risorse da attribuire ai Comuni a compensazione del minor gettito ICI. Anche in questo caso si intravede il disegno unitario e completo del Governo, che punta a fare la propria parte in questo momento di crisi e che credo la stia facendo in maniera efficace. Ho tratteggiato solo due elementi, ma potremmo il Governo ha ben usato lo strumento del disegno di legge sull'assestamento, che peraltro abbiamo visto uno degli strumenti - come direbbero i colleghi sociologi - maggiormente liquidi tra i provvedimenti di finanza pubblica (tanto che diventerà eventuale ove fosse approvata la riforma della contabilità). lo usa però nella maniera più efficace, per avere un altro veicolo idoneo a fronteggiare la crisi e a venire incontro alle necessità soprattutto dei cittadini, ma anche delle imprese e del tessuto produttivo e finanziario nel suo complesso. Così, a mio avviso, va letto il provvedimento e in questo modo mi è parso che siano state inutili tutta una serie di polemiche che hanno

convintamente votare a favore del disegno di legge di assestamento e, naturalmente, anche del rendiconto generale. Per tali ragioni la maggioranza voterà

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1645, nel suo complesso. Colleghi, per cortesia, potete prendere posto?

Dichiaro aperta la votazione.